L'urgenza, già manifestata nei primi giorni del mese di agosto attraverso un'attività di sindacato ispettivo, è necessitata dal fatto che numerose imprese, che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ai sensi della legge n. 388 del 2000, si trovano ad affrontare da alcuni mesi gravissimi problemi economici e finanziari a seguito della comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria della perdita del beneficio fiscale per mancato invio del modello CVS, con relativa richiesta da parte di Equitalia di restituzione del contributo e con eventuale blocco di tutti i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni per importi superiori ai 10.000 euro e fino a concorrenza dell'importo del contributo stesso. Come

questo del giorno in sostanza si invita il Governo a chiarire in termini brevi, attraverso un'interpretazione autentica, limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 62 della della legge n. 289 del 2002, che nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore di dette disposizioni, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002 e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare a quella data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS. Intervengo, signor Presidente, anche per illustrare l'ordine del giorno G3.231, inerente alla legge n. 13 del 1989. Attraverso questo ordine del giorno si vuole impegnare il Governo a stanziare le risorse necessarie affinché 13 del 1989 possa essere adeguatamente rifinanziata, in modo tale da ripristinare quell'importante strumento di concessione ai soggetti diversamente abili dei contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti, finalizzati appunto al miglioramento dei contesti abitativi. Io credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, che abbiamo il dovere morale di garantire la piena dignità delle persone diversamente abili e, soprattutto, l'obbligo costituzionale di rimuovere quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, ma, ancor prima, abbiamo il dovere di dare piena attuazione alle leggi che il Parlamento Non è possibile legiferare, creare aspettative nei cittadini e poi non procedere alla relativa copertura finanziaria, se vogliamo restituire credibilità alla politica e prestigio e autorevolezza alle istituzioni che ci onoriamo di rappresentare per nome e per conto dei cittadini.

Presidente, in merito all'ordine del giorno G3.162 volevo semplicemente ricordare che in sede di esame dell'Atto Senato n. 1209, che reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria è in corso oggi un contenzioso che riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la comunità dell'alta formazione delle accademie e dei conservatori di musica. Questo contenzioso riguarda l'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dall'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativi alla riorganizzazione delle cattedre, contenzioso che ad oggi ha visto diversi interventi della magistratura, che finora hanno bloccato l'operatività di regolamenti non conformi alla legge. legge. Si paventa, quindi, visto l'orientamento che sta ispirando i vari provvedimenti varati nel settore della cultura e dell'università, una posizione che possa portare, prima o poi, ad uno scadimento culturale e professionale del settore delle accademie e dei conservatori di musica qualora si possa porre in atto il tentativo di polverizzare le cattedre e gli insegnamenti, con la conseguente precarizzazione del ruolo degli stessi docenti. Tutto ciò porterebbe anche delle gravi conseguenze all'*iter* formativo degli studenti. Vorrei ricordare, Presidente, che in base alla legge n. 508, attesa dal settore dell'arte italiana, musica e dell'arte in generale, abbiamo ottenuto che il diploma conseguito nei conservatori e nelle accademie avesse valore di laurea a tutti gli effetti, modificando anche il corso formativo degli stessi ragazzi e ragazze che accedevano ai conservatori ed alle accademie, prevedendo quindi prima dell'accesso finale un esame di Stato che riguardava la scuola secondaria. Abbiamo compiuto un'operazione di giustizia, perché nel campo internazionale i nostri giovani, anche se erano direttori di orchestra, non potevano partecipare ai bandi di concorso internazionale perché il diploma conseguito non aveva valore di laurea.

disattesa per lo specifico puntiglio di un direttore generale, che ne fa una questione sua quando questa legge è stata votata

nel solco del dettato della legge, vengano emanati, rendendo giustizia a questo settore dell'alta formazione musicale e artistica. Anche l'ordine

Penso che così come abbiamo effettuato delle operazioni per detrarre dalla denuncia dei redditi le spese per gli animali domestici

per cui un cittadino è libero quando sa scegliere perché ha dentro di sé gli strumenti per poter scegliere: una mente critica e libera che soltanto la cultura può determinare, la capacità di leggere e di leggere con consapevolezza, cercando di comprendere ciò che si legge, nel dettato generale della società ma anche e soprattutto attraverso il libro.

una serie di percorsi e di problemi che sono complessi, ma è anche vero che la cultura di un Paese è tanto più solida quanto più è consolidata attraverso uno sforzo individuale e complessivo della società, ed in particolare della scuola, nell'apprendere attraverso questo strumento che è ancora il libro.

sugli ordini del giorno G3.164 e G3.194. Il primo riguarda tutta la questione del precariato della scuola: spesso infatti sono intervenuta in quest'Aula a sostegno anche di decisioni definitive di questo comparto. Nella scuola italiana insegnano oltre un milione di docenti, di cui 800.000 donne e circa 240.000 precari: il numero esatto dei precari non si conosce ancora, non lo conosce nessuno. Dai dati ministeriali una cosa è certa: solo 700.000 insegnanti possono contare su un contratto a tempo indeterminato. Dei 240.000 assunti lo scorso anno, 22.000 sono stati assunti fino al 31 agosto, 120.000

Due dati sono evidenti tra gli insegnanti italiani: una percentuale molto alta di donne - circa l'81 per cento - e, ovviamente, un'età media che supera abbondantemente i 40 anni. La legge finanziaria del 2006 predisponeva un piano di assunzione di circa 150.000 precari, fino al totale assorbimento delle graduatorie permanenti. Nell'attuare questa disposizione il precedente Governo provvedeva all'assunzione di circa 50.000 precari come prima *tranche*, mentre il ministro Gelmini, all'atto del suo insediamento, tagliava la seconda *tranche* della metà, per cui risultano non ancora immesse in ruolo oltre 75.000 persone. Con l'ordine del giorno, che ho presentato insieme ai colleghi Rusconi, Soliani, Amati ed altri, si predispone il rispetto del piano su un numero che già abitualmente è inquadrato nelle scuole italiane, soprattutto alla luce della decisione di qualche ora fa con cui il ministro Gelmini ha rinviato la riforma delle superiori al 2010. L'altro ordine del giorno, completamente diverso, riguarda il comparto dell'agricoltura, così duramente colpito anche con la pioggia delle ultime ore, e inquadra la crisi della olivicoltura, a causa del calo del prezzo dell'olio extravergine di oliva dovuto alla massiccia importazione dall'estero, alle ingenti giacenze che ingrossano i nostri magazzini e alla lunga siccità estiva ed autunnale che ha colpito intere zone della penisola, soprattutto pugliesi. Tenuto conto che l'olivicoltura pugliese occupa il 54 per cento dell'intera superficie coltivata e che a seguito dell'incontro avvenuto il 17 novembre con il ministro Zaia le categorie hanno richiesto una serie di interventi, come l'immediata liquidazione immediata del premio unico comunitario da parte dell'AGEA, l'attivazione delle misure previdenziali per le calamità e infine l'applicazione del decreto sull'etichettatura di origine delle olive, nell'ordine del giorno si richiede il rispetto di tale impegno da parte del Ministro Ministro e l'immediata esecuzione del programma. l'ordine del giorno G3.165 riguarda i funzionari statali e dell'università che si trovano nelle qualifiche ad esaurimento; quelli che negli anni Settanta venivano reclutati con concorsi severi, nazionali, per soli laureati e, con la normativa allora vigente, percorrevano una carriera che li avrebbe portati ai vertici dell'amministrazione della cosa pubblica, cioè alla dirigenza. Erano figure che garantivano, proprio perché avevano svolto e vinto concorsi nazionali, una serietà di comportamento e di conoscenze. Purtroppo, una serie di norme sopravvenute negli ultimi vent'anni hanno precluso loro di arrivare al vertice della carriera, La legge n. 145 ha risolto in parte questa problematica.

cento imposta dall'articolo 5 della legge n. 145 del 2002, che pertanto restringe il campo di applicazione ad un numero veramente esiguo di aventi diritto. L'ordine del giorno fa riferimento alle università

Presidente, onorevoli colleghi, questo è un tema di straordinaria attualità ed è anche un indice della civiltà di questo Paese:

Commissione sulle morti bianche e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, non solo per creare una condizione di prevenzione ma anche per creare una responsabilità diffusa, perché un Paese civile non si può permettere un milione di infortuni e 1.200 morti sul

fra tutti i livelli istituzionali si possa realizzare un'azione di prevenzione e di incentivo per tentare di eliminare questa piaga e questa tragedia, per riportare questo Paese in una condizione di civiltà.

in modo da assicurare la parità di condizioni tra le lavoratrici subordinate e quelle parasubordinate nell'accesso ai trattamenti di maternità, garantendo a queste ultime l'automatismo della prestazioni.

secondo il rapporto di monitoraggio del ministero del lavoro del 2008, appena il 31 per cento dei disoccupati è coperto nel nostro Paese da un ammortizzatore sociale; Le stime ad oggi disponibili in merito a quelli che potrebbero essere gli effetti della crisi economica riportano cifre preoccupanti: 2 milioni potrebbero essere i disoccupati negli anni 2009-2010, 300.000 i precari che già dalla fine di quest'anno potrebbero vedere a rischio il loro contratto o comunque trovarsi in una situazione di non occupazione, tutti senza una rete di protezione sociale.

degli ammortizzatori sociali; una riforma che doveva rivedere completamente questa materia, eliminando la divisione tra garantiti e non garantiti prevedeva testualmente la graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati, senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione d'impresa e tipologia dei contratti di lavoro. Bene (o forse dovremmo dire male), purtroppo le misure presentate dal Governo per contrastare la grave crisi economica in realtà prevedono semplicemente di proseguire sulla strada fino ad oggi percorsa, lasciando quindi inalterato il sistema attuale, con la suddivisione tra i garantiti e i non garantiti e in particolar modo con la decisione di finanziare ulteriormente la cassa integrazione straordinaria. Ricordo

ben 120 miliardi di euro, senza che un solo posto di lavoro venisse salvato. Di fatto, probabilmente dovremmo ripensare tutto, ma dovremmo farlo anche perché c'è una delega al Governo che va proprio in questa direzione.

30 giugno del 2009, alla riforma integrale degli ammortizzatori sociali nella direzione della legge delega e, quindi, anche all'abolizione della Cassa integrazione straordinaria. In sostanza, il sostegno deve andare ai lavoratori che perdono il lavoro,

un aiuto alle imprese che spesso sono decotte: è inutile ricordare il caso di Alitalia.

Badate che il ceto medio-basso, ossia chi è in difficoltà in Italia, guarda al sistema sanitario del nostro Paese come ad un momento di sicurezza. In una società complessa come la nostra, il sistema sanitario è un punto di riferimento di forte solidarietà nel Paese. Tagliare la sanità in questo momento non significa renderla più efficiente, ma semplicemente tagliare la solidarietà, e non penso che questo Governo voglia con una mano seminare speranza e con l'altra preoccupazione. Questi tagli alla sanità destano viva preoccupazione. Siamo convinti che il sistema sanitario nazionale, che ha 30 anni di vita, sia al momento un buon sistema perché garantisce a tutti la certezza e l'accesso alle cure, con la modalità universalistica e solidaristica; tagli è sbagliato, soprattutto perché si deprime al basso e non si mette in evidenza la qualità che esso esprime. Ci sono grandi disparità nel Paese tra Nord e Sud e dobbiamo sicuramente razionalizzare il sistema, ma non è tagliando in modo lineare che avviene la razionalizzazione. Ci sono altre modalità che, tra l'altro, abbiamo condiviso all'interno della Commissione sanità con il Governo stesso, che ha accolto un ordine del giorno per l'incremento degli investimenti sull'edilizia ospedaliera e anche su alcuni meccanismi di miglioramento della remunerazione della spesa sanitaria che affianchi alla quantità anche la qualità.

che ci impegniamo ad accompagnare ad un meccanismo di razionalizzazione e di recupero di efficienza all'interno della spesa sanitaria stessa. Chiediamo un segnale di disponibilità che penso sia

all'ordine del giorno G3.198 sia stata posta la mia firma; chiedo quindi che venga cancellata. Inoltre richiamo brevemente l'attenzione del rappresentante del Governo e del relatore sui contenuti dell'ordine del giorno G3.130. Il documento tratta dell'annosa questione riguardante i cittadini italiani autoctoni di Istria, Fiume e Dalmazia che, a seguito degli eventi bellici della seconda guerra mondiale, furono costretti ad abbandonare quei luoghi. Nel merito voglio sottolineare che nei documenti finanziari alla nostra attenzione subiscono una consistente decurtazione i fondi assegnati per l'applicazione delle disposizioni normative in materia di indennizzi ai cittadini italiani e alle imprese operanti nei territori della ex Jugoslavia. Tenuto conto però, signor Presidente, che rimangono ancora da evadere numerose richieste si chiede al Governo di voler stanziare, con il prossimo provvedimento finanziario, tutte le risorse necessarie a garantire il riconoscimento di un equo e definitivo indennizzo ai richiedenti ancora in attesa della giusta liquidazione. Spero nell'accoglimento dell'ordine del giorno in

mi pare che l'andamento del dibattito in Aula e delle votazioni potrebbe consentire, diversamente da quanto si era convenuto nella Conferenza dei Capigruppo

di bilancio e finanziaria nel corso della seduta odierna. Credo vi siano le condizioni perché questo possa avvenire in parziale modifica del calendario

e di svolgere qualche breve considerazione su questo tema. Signor Presidente, non ci opponiamo. La richiesta del senatore Gasparri ci è arrivata anche dal anche dal Capogruppo della Lega Nord; ci è pervenuta in modo cortese e soprattutto in modo motivato. È stato posto il problema che riguardava le difficoltà legate al sistema dei trasporti nazionali nella giornata di domani; questo problema riguarda molti senatori non solo della maggioranza, ma anche dell'opposizione. Signor Presidente, noi non facciamo dispetti, non facciamo prepotenze; avevamo interesse a che la seduta di domani vedesse svolgere le dichiarazioni di voto ed il voto su un provvedimento così importante, ma riteniamo motivata la richiesta, per cui diamo il nostro assenso. sottolineare anche qual è il limite di questo assenso. Noi accediamo al fatto che venga modificato il calendario dei lavori dell'Aula, ma non stiamo rinunciando ai nostri diritti; non stiamo rinunciando al tempo che abbiamo a disposizione, perché è stato così determinato, e non stiamo rinunciando a utilizzare il Regolamento. Lo voglio ricordare oggi perché due settimane fa siamo stati, siamo stati, invece, indicati come prepotenti per aver voluto usare gli strumenti che il Regolamento ci consentiva di usare.

ma non marginale episodio svoltosi ieri mattina in quest'Aula. L'ho seguito da lontano, perché dal mio banco non potevo apprezzare le circostanze nel loro dettaglio, però ho visto molto chiaramente la senatrice Mongiello, senatrice Segretario dell'Assemblea, circondata da molti colleghi senatori che le urlavano in faccia. Ora, voglio dire questo in modo molto chiaro e con molto rispetto: io credo che tutta l'Assemblea debba rispettare i Presidenti dei Gruppi parlamentari e quindi concordo con la richiesta fatta ieri in Aula dal senatore Quagliariello affinché tale rispetto venga garantito. Tuttavia, un rispetto ancora maggiore ai senatori Segretari d'Aula, come lo dobbiamo al Presidente dell'Assemblea, perché svolgono un compito molto ingrato e molto difficile, che noi dovremmo cercare di agevolare. credo - mi rivolgo al mio Gruppo, ma anche alla maggioranza che vedo meglio perché l'ho di fronte durante le votazioni - che sia dignitoso per noi alzarsi in piedi per impedire che si veda la luce nostro quando si vota. Non credo che sia dignitoso non sedersi al nostro posto in modo che sia difficile controllare. Io credo - e mi rifaccio alle richieste da lei più volte ripetute, Presidente - che se noi durante le votazioni fossimo

Presidente, noi siamo davanti a un momento molto delicato della legislatura. Abbiamo sul tappeto il federalismo fiscale e il tema della giustizia. Io vorrei sapere - questo ha a che fare con i rapporti tra maggioranza e opposizione e ha a che fare con la nostra attività legislativa - se la maggioranza, e per essa il Presidente del Consiglio, intende

l'argomento è molto serio. Ci stiamo dicendo da più legislature che le grandi riforme si fanno insieme. Ieri abbiamo sentito il Presidente del Consiglio ricordarci che addirittura la Costituzione si può cambiare da soli! Vorrei sapere, per potermi personalmente regolare nei rapporti politici con la maggioranza, se questa linea viene confermata e se noi dell'opposizione, sul federalismo fiscale, dobbiamo atteggiarci

il ministro Bossi ha indicato al Presidente del Consiglio. Infatti, con una dichiarazione che trasuda saggezza, gli ha detto e insegnato che le questioni personali non devono diventare questioni politiche. Signor Presidente, affido a lei

L'ho fatto pubblicamente, anche in occasione di riunioni istituzionali, e in ogni occasione che mi è stata data, sia privata che pubblica. Tra l'altro, l'adesione odierna alla richiesta della maggioranza di concludere i nostri lavori

darvi merito, perché è proprio di un'opposizione responsabile assumere atteggiamenti e toni quali quelli che sono stati assunti fino ad oggi in quest'Aula da parte dell'opposizione. da lei posto, presidente Zanda, ho registrato, come lei, alcune dichiarazioni che hanno costituito un momento di forte dibattito politico. Sono e rimango dell'idea che per le riforme occorra lavorare quotidianamente, per trovare il massimo del consenso.

Questa dichiarazione, ove dovesse essermi confermata, va nel senso di un'apertura ad un confronto, quanto meno secondo la stessa dichiarazione del Presidente del Consiglio.

si possa trovare un dialogo anche sulle questioni che riguardano la vita dei cittadini perché finora su questioni importanti, come la

limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002,

2), accolti come raccomandazione,

il Governo: al fine di sostenere i settori produttivi in recessione e promuovere il *made in Italy* a valutare l'opportunità di prevedere interventi ed eventuali finanziamenti finalizzati a potenziare la vocazione internazionale,

l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Colgo l'occasione per ringraziare il Senato per l'impegno che sta profondendo nell'esame dei documenti finanziari.

rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, a proposito di questo emendamento, che ritiro, constatata la posizione del relatore e del Governo, chiedere che fosse accolto come ordine del giorno, con una modifica, onorevole Sottosegretario, che sostanzialmente è una raccomandazione: quella per cui il Ministero competente Ministero per i beni e le attività culturali - in applicazione dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, rimodulando le risorse, tenga conto della necessità - che si riferisce alla condizione

voglio fare una brevissima dichiarazione di voto perché credo sia utile per l'Aula conoscere il contenuto di questo emendamento e soprattutto sapere che cosa sta accadendo nel mondo della montagna italiana. L'anno scorso, con la legge finanziaria, noi facemmo una riforma seria, indicando alle Regioni obiettivi di riduzione, di eliminazione di storture e di sprechi, anche sull'onda delle polemiche che c'erano state su questa materia. Ebbene, a distanza di un anno, 13 Regioni su 15 si sono adeguate a quella normativa. Le comunità montane si ridurranno da 330 a 170; il peso degli organismi politici, in termini numerici, si ridurrà del 60 per cento a riforme già approvate;

risultati importanti che sono andati esattamente nella direzione auspicata dalla norma che licenziammo l'anno scorso. il Governo e la maggioranza hanno ulteriormente ridotto, non tenendo conto di questo sforzo riformatore molto serio, anche il fondo ordinario

La maggioranza aveva affermato nel programma elettorale di voler abrogare le comunità montane ma ha scelto, invece, di asfissiarle finanziariamente con il rischio che le stesse

**Il Senato non approva.**

perché è volto a promuovere un'attività, come ho avuto modo di dire questa mattina, diretta a sollevare le popolazioni civili dai patimenti che molto spesso queste devono vivere anche al di là

L'Italia è - come afferma il professor Gallino - «uno dei Paesi più diseguali al mondo». In pari tempo è quello che negli ultimi dieci anni ha un tasso di crescita pari a meno della metà della media europea. È il Paese che cresce meno, che ha un tasso di povertà minorile tra i più alti dell'Occidente, il tasso demografico più basso e un numero di famiglie povere elevato tra quelle monoparentali o con figli. L'Italia ha insufficienti servizi e al Sud sono quasi assenti; inoltre, ha il tasso di occupazione femminile - come hanno rilevato molte colleghe - molto al di sotto della media europea. Questo quadro non è il frutto del caso (ed anche oggi l'UNICEF ci ricorda che l'Italia è agli ultimi posti nell'OCSE per servizi all'infanzia e a moderne politiche per le famiglie), bensì di una visione arretrata ed inadeguata a governare i processi di cambiamento in atto nelle famiglie, nella società e nell'economia. Le misure proposte dal Governo aggravano ulteriormente questo quadro. Era necessario uno scatto, c'era bisogno di un'azione straordinaria. Perlomeno si potevano mantenere i fondi deliberati dal Governo Prodi: il fondo sociale, quello delle famiglie, dell'infanzia e adolescenza, sulla non autosufficienza, sull'immigrazione, sulle politiche giovanili, sul piano decennale sui nidi. All'opposto non c'è stata alcuna azione straordinaria ed anzi si tagliano tutti i fondi per 660 milioni e contemporaneamente si sottraggono miliardi agli enti locali, che così non possono più garantire l'erogazione dei servizi e l'aiuto alle persone e alle famiglie in difficoltà. In Europa, in molti Paesi, ci si confronta con la globalizzazione, non arretrando rispetto al modello sociale europeo, che è quello di una società aperta, che rilancia la sua sfida su un'idea per cui è, sì, scandalosa la povertà, ma ancor più lo è la mancanza di eguali opportunità di vita. In Europa c'è un altro approccio alla spesa sociale; c'è la consapevolezza che una quota crescente di spesa sociale dovrà avere carattere di investimento, che la spesa per i servizi sociali per attivare le risorse personali e familiari contro i rischi può comportare dividendi nel lungo periodo per gli individui e per la società nel suo complesso. La migliore assicurazione contro le paure e i rischi legati alla stessa globalizzazione è un *welfare* attivo che sostiene chi fronteggia il rischio, che scommette sul capitale umano di ognuno, sulle famiglie, che contrasta le disuguaglianze e ridistribuisce *chance* di vita. Certo, è una concezione che presuppone dei valori, ma chi può dire che i valori siano antinomici ai vincoli di bilancio o frenino la competitività? Nella storia del *welfare* europeo, nei Paesi più forti, la cittadinanza è sempre più legata all'eguaglianza delle opportunità, oltre che all'azione di protezione sociale dalle avversità. Ha prevalso in questi Paesi un'interpretazione universalistica dei diritti sociali con un'estesa offerta di servizi pubblici. La redistribuzione delle *chance* diventa allora sia un valore fondamentale per società democratiche, non oligarchiche, ma anche un fattore fondamentale di sviluppo. Colleghe e colleghi, senza gli ultimi non si diventa primi; questo hanno capito i Paesi che oggi guidano lo sviluppo e che investono sulle capacità di ognuno e sui bambini, su tutti i bambini, sostenendo anche le loro famiglie, perché insieme all'affetto possano dare loro il sostegno per sviluppare tutte le loro capacità. Le famiglie vanno difese a partire, tenendo presente il reddito, da quelle monoparentali e da quelle con più figli. Almeno ci si ripensi e si accolgano alcuni degli emendamenti presentati,

Penso che non si esca dalla crisi ripiegando e questo provvedimento è anche un ripiegamento; se ne esce contrastando con rigore gli sprechi e l'evasione fiscale, premiando il merito e riaprendo quindi la via a chi può aver fiducia in un Paese che non lo lasci solo, che investa sulle sue capacità e risorse, e lo metta in grado di fronteggiare i rischi e cogliere tutte le opportunità, insomma di tenere sotto controllo la paura e aprirsi alla speranza.

gli studenti universitari fuori sede che arrivano nelle grandi città e, naturalmente, non riescono a trovare un alloggio adeguato né case degli studenti e delle studentesse che possano accoglierli per fare loro svolgere un'attività di studio tranquilla. Sono sempre a carico dei genitori e alcuni devono anche lavorare. Mi rendo conto che in questa finanziaria - e chiudo, signor Presidente - c'è un Ministro che ricorda tanto il principe di Valacchia, duca di Amlas e Fagaras e cavaliere del Sacro ordine del drago. Ci riferiamo naturalmente al conte Dracula che ha rastrellato ovunque e ha aumentato anche la pressione fiscale; però, 7 milioni di euro per aiutare gli studenti

impegna il Governo a far rispettare una legge dello Stato, che questo Parlamento ha votato e che l'INPS invece, con delle circolari, quindi con norme di rango legislativo assolutamente inferiore, si ostina ad osteggiare e a

Presidente, non vorrei che di questo passo saremmo costretti a fare una colletta tra di noi per il Governo.

Il Ministro dell'economia tira fuori dal capitolo relativo al dissesto idrogeologico della Sicilia e della Calabria 151 milioni di euro,

Presidente, facciamo così: il Senato voti se vuole impegnare il Governo a ripristinare questi fondi oppure no!

Quest'ultima è sin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e, quindi, a riferire all'Assemblea. Sospendo pertanto la

Colleghi, prima di riprendere con i successivi adempimenti i nostri lavori, preciso, in relazione a richieste avanzate da onorevoli colleghi, che la decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo di concentrare le dichiarazioni di voto sul complesso dei documenti finanziari nella fase finale, e cioè subito prima del voto del bilancio dello Stato, è conforme ad una prassi della nostra Assemblea che vede spesso i Gruppi pronunziarsi proprio prima del momento conclusivo della complessa procedura di esame della finanziaria e del bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del sottosegretario Vegas, ha presentato la Seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 tendente ad introdurre nel testo del disegno di legge del bilancio e nelle annesse tabelle le modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della legge finanziaria. Tale Nota è stata deferita alla 5a Commissione permanente. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Saia,

è stata predisposta al fine di recepire gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica al disegno di legge finanziaria 2009 e al progetto di bilancio, in sede di seconda lettura del testo approvato dalla Camera dei deputati, nel quale erano già considerati, mediante apposita Nota di variazioni, gli effetti della prima lettura. È da porre in evidenza che gli emendamenti al disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 e al progetto di bilancio per il triennio 2009-2011, in esito alla valutazione degli effetti finanziari dai medesimi determinati, riflessi nella presente Nota di variazioni, non comportano, rispetto agli obiettivi prefissati nella manovra, effetti peggiorativi dei saldi di finanza pubblica. Le implicazioni finanziarie, contenute nella Seconda Nota di variazioni, comportano modifiche: ai quadri generali riassuntivi per l'anno 2009 in termini di competenza e di cassa; al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009-2011 in termini di competenza; agli Stati di previsione della spesa di taluni Ministeri (tabelle nn. 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 12). Inoltre, un migliore apprezzamento delle variazioni medesime e dei relativi effetti sui saldi e sui vari documenti del bilancio di previsione si ricava dagli elaborati relativi ai quadri di sintesi dei dati del bilancio per l'anno 2009 in termini di competenza e di cassa al netto delle regolazioni contabile e debitorie (allegati nn. 1 e 2).

due problemi che riguardano la significatività del bilancio a questo punto al nostro esame. Naturalmente, la Nota di variazioni corrisponde alle esigenze sotto il profilo tecnico, nel senso che trasferisce al bilancio le variazioni intervenute nella legge finanziaria così come l'abbiamo approvata qualche minuto fa. Sotto il profilo, quindi, della specificità e delle caratteristiche tecniche della Nota di variazione non vi è nessuna questione. Tuttavia, nel corso del dibattito ho sollevato un problema relativo alla significatività del bilancio per quello che riguarda il Fondo per le aree sottoutilizzate. Adesso, richiamando brevemente quell'argomento, voglio aggiungere il problema rappresentato dalla significatività del bilancio che il Senato della Repubblica si appresta a votare circa il suo carattere, o politicamente o tecnicamente, poco veritiero - per usare un'espressione eufemistica - a proposito del Ministero della pubblica istruzione. Signor Presidente, oggi il Ministro della pubblica istruzione ha sostanzialmente dichiarato due cose. Ha detto, in primo luogo, che il cosiddetto maestro prevalente (evoluzione dell'idea del maestro unico nella scuola primaria) verrà introdotto esclusivamente a richiesta delle famiglie. Questa è la prima cosa che ha detto oggi il Ministro al termine - mi pare - di un incontro con le parti sociali. Una seconda affermazione fatta dal Ministro è che gli interventi di ristrutturazione sulla scuola secondaria superiore saranno rimandati ad un anno successivo (dal 2009 al 2010). Ora, signor Ministro, sotto il profilo politico noi prendiamo atto positivamente dell'una e dell'altra affermazione. Non avrebbe senso parlarne in questa sede se non ci fosse un problema nel rapporto tra queste affermazioni e il bilancio che stiamo per approvare. Signor Ministro, i risparmi recati sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione dal decreto n. 112 e dal successivo decreto cosiddetto Gelmini sono ovviamente incorporati nel bilancio a legislazione vigente, cioè quello che siamo oggi chiamati ad approvare, non essendo intervenuta per questo aspetto alcuna scelta nella legge finanziaria che mitiga i tagli operati legittimamente sul piano politico - ci mancherebbe - e legittimamente sul piano tecnico con quelle decisioni.

ma allora il bilancio di questo Ministero è tecnicamente non veritiero; oppure - come io penso che sia - il Ministro ha torto e la legislazione vigente non consente al Ministro stesso di fare quello che oggi il Ministro ha annunciato.

la seguente: il bilancio a legislazione vigente è quello che deriva dall'applicazione puntuale e corretta del decreto n. 112 e del successivo decreto Gelmini; però, il bilancio a legislazione vigente è tecnicamente corretto per quello che riguarda il Ministero, ma questo mette in mora politicamente il Ministro che non potrà fare le cose che oggi ha enunciato. In secondo luogo, insisto, il bilancio a legislazione vigente prevede un'appostazione al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) che non è tecnicamente corrispondente all'utilizzo di quel fondo come mezzo di copertura per decreti in vigore, quindi per coprire coprire legislazione vigente. Questo significa, signor Presidente, che almeno per la parte relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, il bilancio che ci apprestiamo a votare è tecnicamente falso. *(Applausi dai

fotogramma che passa in un dato momento. In quel dato momento non può passare altro che ciò che è già registrato dalla legislazione vigente, mentre le evoluzioni successive si registreranno a bilancio in un momento successivo. La stessa cosa vale per il Fondo aree sottoutilizzate, perché anche in questo caso, come è sempre stata prassi in caso di presentazione della Nota di variazioni, non si tiene conto di quanto si va realizzando con la legislazione, ma si registrano esclusivamente le modifiche che, attraverso il disegno di legge finanziaria, vanno riportate a bilancio.

signori del Governo, colleghi, la mia sarà una dichiarazione breve, non soltanto perché

in un rito inutile, nel quale lo spazio emendativo è stato sostanzialmente impedito, che manca di forza propositiva

soprattutto tra chi si aspetta che questo Governo abbia equilibrio nel considerare le diverse esigenze ormai diventate stringenti, soprattutto nell'area del Mezzogiorno, che

soprattutto per forze politiche che, pur volendo sostenere il Governo con convinzione, hanno difficoltà ad interloquire nella fase di predisposizione dei provvedimenti nel Consiglio dei ministri o, comunque, nell'ambito di un sistema di maggioranza che assicura un'interlocuzione reale.

risolvere alcune ferite aperte, alcuni torti che erano stati ampiamente riconosciuti dal Governo con rassicurazioni verbali, formali sempre più frequenti, ma sempre più inutili.

il voto formale di approvazione a questo provvedimento, ma consentitemi - questa volta scelgo un altro aggettivo - è un voto formale che ritengo assolutamente inutile. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, l'esame del disegno di legge finanziaria si sta svolgendo nel pieno di una tempesta finanziaria che, come ha ricordato il Governatore della Banca d'Italia si è già scaricata sull'economia reale attivando un circolo vizioso dal quale ancora non si vede una via di uscita. Siamo in un momento, signor Presidente, di grande confusione e precarietà e chi ostenta, come ha ostentato, grande sicurezza dovrà comunque subire una verifica nel tempo. D'altra parte, la mancanza di fiducia si sta espandendo: da un lato le imprese sono costrette a tagliare molti piani di investimento e risentono della stretta, dall'altro i consumi ristagnano e tendono ad indebolirsi ulteriormente. Alla drammatica congiuntura si somma per il nostro Paese una specifica difficoltà competitiva tutta interna al nostro sistema produttivo ed amministrativo. E qual è l'approccio che ci propone questa finanziaria? Contempla una grande unica misura: non aumentare la spesa e poco altro. L'errore della manovra economica di luglio appare oggi ancora più evidente, clamorosa. Un' assenza di lungimiranza ha caratterizzato quelle scelte. Eppure già in occasione del dibattito parlamentare era stato avvertito il Governo che bisognava cambiare strada. La crisi infatti, anche se non nelle dimensioni attuali, era già conosciuta ed il taglio dell'ICI, da solo, ha sottratto alle casse dello Stato più di 3 miliardi di euro e Dio sa quanto oggi sarebbe utile A questa emergenza va aggiunto un altro elemento cruciale rappresentato dal rischio - è questo il grande pericolo che si va concretizzando - che molte persone nei prossimi mesi perderanno il loro lavoro. Ci sembrava necessario, che in questa situazione il Governo rivedesse la scelta di concentrare tutta l'azione economico-finanziaria nel decreto-legge n. 112. Quello strumento e quella impostazione sono invero superati dai fatti. Questa finanziaria, invece, non torna indietro rispetto ai tagli della spesa per investimenti, non li rimodella né li riduce. Alla luce delle nuove emergenze, in questo modo non si tagliano gli sprechi, sui quali è opportuno continuare ad intervenire, ma che vanno distinti dagli interventi che tagliano potenzialità di sviluppo. L'esempio di gestione inconsulta del Patto di stabilità, incapace di distinguere tra enti locali virtuosi e viziosi, penalizzati tutti addirittura allo stesso modo, è clamoroso. Io stesso ho sottolineato - ma devo ammettere che sono stato ascoltato - il paradosso della Valle d'Aosta che ha più entrate di quello che può spendere e ha un avanzo di bilancio consistente che non può spendere. Ma a parte un ascolto corretto e condiviso da molti, non c'è stato molto di più. In sostanza, la caratteristica di questo disegno di legge non è data da quello che c'è, quanto piuttosto da quello che manca, da quello che non c'è. Per la sanità, mi permetto di dire, non è solo una questione di finanziamenti. Si può risparmiare anche modificando i modelli, i mansionari. Siamo ormai sempre più convinti che sia necessaria una manutenzione della legge sul sistema sanitario nazionale. Senza ulteriori cambiamenti In questa discussione sulla finanziaria abbiamo provato ad agire su alcuni aspetti che potrebbero avere un positivo impatto sui cittadini. Abbiamo presentato emendamenti contenenti misure relative alla la vera dimenticata da questa manovra. Le nostre proposte vanno tutte verso l'obiettivo di garantire detrazioni alle famiglie con figli a carico, emendamenti che, il più delle volte, non sono stati Ricordiamo che la nostra proposta era di 1.200 euro per ogni famiglia con un figlio, cui sommare per ogni altro figlio. Ciò avrebbe comportato un costo di 6 miliardi di euro: il salvataggio di Alitalia è costato molto di più! Signor Presidente, mi rivolgo al Governo ed alla maggioranza, scevro da ogni accento polemico, perché, come ci insegnano le grandi democrazie, ci sono momenti nei quali bisogna far prevalere l'interesse generale alle legittime convenienze di parte. E allora, prendete sul serio quanto vi diciamo, cioè che è necessario ed urgente cambiare linea; prendeteci sul serio quando vi diciamo che dobbiamo estendere la copertura assicurativa dal rischio di disoccupazione, per creare un ponte che ci consenta di attraversare la fase più acuta della crisi, riducendo il rischio che l'incalzare della stessa provochi un aumento della disoccupazione che blocchi il processo di allargamento della base occupazionale. In caso contrario, infatti, la ripercussione sulle condizioni sociali di vasti strati di famiglie sarà drammatica, ben più seria dell'obiettivo - oggi ancora perseguibile - di rilanciare la loro capacità di consumo. Concludo riconoscendo che questo Governo e questa maggioranza avevano iniziato a giocare all'attacco - è vero - facendo anche scelte coraggiose e giuste; ma ora siete lì a mantenere posizioni,

tutto il deliberato di questo mese di fine d'anno, argomento della finanziaria, lo avete inserito in altri decreti che sono stati approvati e che verranno approvati.

me lo permettano gli amici del Governo perché credo che da lì sia venuto l'ordine - concerne l'inammissibilità. Si è giocato molto sull'inammissibilità di alcuni emendamenti. È stata utilizzata come un'arma per bloccare anche la discussione in Aula. Tanti provvedimenti presentati dagli amici dell'opposizione, anche da voi della maggioranza: argomenti validi, provvedimenti validissimi, riconosciuti nelle Commissioni sono stati

a strumentalizzare il terremoto! Avevamo presentato degli emendamenti, signor Sottosegretario; avevamo detto che il Governo doveva farli propri, che anche il

Avete negato ogni modifica - ve lo dobbiamo dire - ad eccezione di tre piccole cose: sul Patto di stabilità, sull'area di confine per accontentare alcuni partiti amici, che altrimenti forse non vi votavano. Per non dire della scuola privata! Vi hanno pregato nella Commissione:

Ci è voluto l'intervento esterno della gerarchia ecclesiastica per far rimettere questi soldi. Con tutto il rispetto da cattolico praticante che ho per la gerarchia ecclesiastica, credo che il Parlamento non doveva subire questa onta. E credo che

Allora, amici, per accelerare le cose, ve lo dico in via ufficiale: anche se veniamo offesi giornalmente (ieri ci sono state ripetute offese), anche se noi dell'Italia dei Valori veniamo indicati come forza eversiva, vi diciamo che di fronte ai problemi seri della nostra gente e della nostra Nazione noi vogliamo collaborare. collaborare e diamo la nostra disponibilità totale, come forza di opposizione, ma certamente non vogliamo più ricevere insulti e dichiarazioni di autosufficienza da parte vostra; in questi giorni le abbiamo sentite spesso, anche da parte del *leader* della maggioranza: «Se volete, volete; se no andiamo avanti lo stesso». In certi periodi

vi ho detto l'altra volta di rassegnarvi perché noi dell'Italia dei Valori non siamo un incidente della storia degli ultimi dieci anni. Vi dovete rassegnare, di qua e di là. Siamo una forza politica e la gente guarda a noi; ci meravigliamo pure di certi consensi e di certi dati e qualcuno ci deve sopportare. Vi diciamo

chi vuole veramente vedere nel federalismo un mezzo per cambiare la nostra Italia. Vogliamo lavorare insieme, ma reagiremo con forza contro chi vuole farci diventare una forza da escludere. Ci siamo,

in raggruppamenti più grandi, in base alle leggi elettorali che saranno approvate, ma intendiamo anche noi servire il Paese e aiutare questa Italia a uscire dalla crisi. Questa finanziaria merita un secco no perché non va in quella direzione.

vorrei fare una premessa importante. Ci dimentichiamo spesso che se siamo qui serenamente a ragionare di questa legge finanziaria è perché il Governo ed il ministro Tremonti hanno avuto l'intuizione di anticipare a luglio il grosso del lavoro e la fissazione dei saldi; altrimenti oggi saremmo in una situazione ben più complicata e complessa. Ciò va rimarcato e ricordato. Ciò detto, in questa snella manovra finanziaria non c'è anzitutto il solito assalto alla diligenza, ed anche questo ricordiamolo. Nella prima finanziaria Prodi le spese sono aumentate di 3 miliardi nella seconda addirittura di 4,5 miliardi di euro: 7,5 miliardi di euro di spese in più proprio causate dall'assalto alla diligenza. Questo per chiarezza ce lo dobbiamo ricordare. Prima il collega Morando faceva un'allusione all'eventuale irregolarità del bilancio. il presidente Baldassarri lo ha ben evidenziato più volte - i tesoretti nascosti sotto il tappeto? Quello sì che era un falso in bilancio! Ma me ne ricordo un altro molto più interessante. Si parla tanto di pressione fiscale:

Così come non è serio l'assalto alla diligenza in una situazione come questa, di oggettiva grave crisi. Dobbiamo però guardare anche in positivo; e iniziamo a farlo con due considerazioni di fondo. Abbiamo tutti una grossa opportunità che, paradossalmente, è proprio l'enorme debito pubblico e l'enorme spesa pubblica. Se iniziamo ad aggredire in maniera seria e convinta la spesa pubblica, che è assolutamente fuori da ogni logica,

punto fondamentale, perché altrimenti oltre alla crescita della disoccupazione, normale in una situazione come quella attuale, avremmo avuto la chiusura

gli investimenti, si è fatto quello che si è potuto fare. La modifica del Patto di stabilità a tassi invariati, comunque, consente di attivare gli investimenti dei Comuni e ciò nella situazione attuale è molto positivo. Il CIPE, il Governo, farà

- che la Lega ha voluto particolarmente è l'intervento e il rifinanziamento del Fondo per le aree al confine con le Regioni a Statuto speciale. Un'operazione - siamo noi della Lega i primi

dove c'è grasso che cola, dove ci sono gli sprechi; si responsabilizza. Abbiamo una grande occasione: l'enorme spesa pubblica. Se riusciamo, insieme, a realizzare questa grande riforma, otterremo un beneficio per tutti: quello di tagliare molto la spesa pubblica e, finalmente, le tasse.

la lunghissima sessione parlamentare di bilancio, apertasi con il Documento di programmazione economico-finanziaria e con il decreto di giugno-luglio e proseguita con l'emanazione di numerosi decreti che ne correggono questo o quell'aspetto, fino al decreto n. 185 in discussione in questo momento alla Camera, sta per chiudersi senza che sia stata fornita dal Governo una risposta almeno chiara, se non convincente, alla seguente domanda: qual è la ragione per la quale il Governo italiano, unico in Europa e nel mondo occidentale, si rifiuta di usare anche la politica di bilancio per per fare fronte alla recessione che già si dimostra pesantissima e che si annuncia molto lunga, purtroppo? Riferendoci ai grandi filoni della teoria economica, le risposte a questa domanda possono essere due. La prima è quella del liberismo puro (il nostro Ministro dell'economia forse lo chiamerebbe fanatismo mercatista): i fattori di soluzione della crisi - così vogliono i liberisti puri - saranno prodotti dalla recessione stessa e nella recessione stessa. È vero che l'aggiustamento e il riequilibrio avranno costi sociali pesanti - licenziamenti, fallimenti di imprese, caduta del reddito - ma essi saranno mitigati dalla forte riduzione dei prezzi e dalla caduta del costo del danaro, che contribuiranno a migliorare progressivamente la domanda sia dal lato dei consumi, sia dal lato degli investimenti, e comunque - concludono i fanatici mercatisti per continuare con l'immagine che piace al Ministro se si intervenisse con politiche di bilancio espansive non si farebbe che rallentare il ritmo dell'aggiustamento aggravandone, lungi dal mitigare, i costi sociali. La seconda risposta è più ritagliata invece sullo specifico italiano: le politiche di bilancio espansive sono certamente raccomandabili - vuole questo orientamento anche di tipo teorico - quando si tratta di contrastare una forte recessione, ma attenzione, esse devono essere rese compatibili con la stabilità finanziaria di lungo periodo; quindi per l'Italia conclude questo orientamento troppo incombente il rischio di peggiorare il merito di credito del Paese con conseguenze insostenibili sulla spesa per interessi. La prima risposta non viene sposata dal Governo Berlusconi. Al di là della sua improbabile coerenza con libri e suggestioni colbertisti e neostatalisti, essa è infatti abissalmente lontana dalla cultura politica di una coalizione di forze che pratica da sempre (e più di recente, per la verità, predica anche un po' più apertamente) politiche ostili all'apertura dei mercati chiusi, esalta l'italianità come valore da difendere ad ogni costo (anche quando l'erario e l'interesse nazionale ne risultano gravemente danneggiati), rinnova pubbliche concessioni per legge, sospende *sine die* normative *antitrust* in settori strategici, aumenta di due punti di prodotto interno lordo in cinque anni la spesa corrente primaria. Insomma, cari colleghi, la signora Thatcher, che da tempo, grazie al New Labour, non abita più al numero 10 di Downing Street, non si è certo trasferita nemmeno in spirito a Palazzo Chigi. Resta allora la seconda risposta, che io riassumo con la posizione «vorrei ma non posso». con l'anomalia indiscussa dei conti pubblici italiani l'anomalia del suo orientamento politico in chiave di politiche di bilancio, un'anomalia che è tale, insisto su questo punto, nell'intero Occidente. Non c'è nessun Governo occidentale che abbia una politica di bilancio ispirata all'orientamento che voi state facendo ostentatamente e ostinatamente vostro. Un tentativo, questo del Governo, del quale la nostra proposta alternativa ha dimostrato l'intrinseca debolezza. Noi non vi abbiamo proposto, signori del Governo, di abbandonare il sentiero della stabilità, né vi abbiamo proposto di abbandonare l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2012-2013: avremmo, se avessimo fatto questo, tradito gli interessi del Paese e avremmo tradito noi stessi, visto che siamo stati noi, non voi, a guidare lo sforzo per conquistarlo quel sentiero. Noi vi abbiamo proposto un'altra strada: nel 2009, abbiamo detto, un peggioramento di un punto di PIL nel rapporto indebitamento netto-prodotto, per usare più di 15 miliardi di euro in misure di contrasto al ciclo negativo e subito, contemporaneamente, le misure legislative ed amministrative che consentono di garantire ai mercati finanziari il permanere della nostra finanza pubblica in un'area di stabilità nel 2010, 2011, 2012. Ieri sono stati pubblicati i dati drammatici della produzione industriale in Italia. Il nostro è un Paese manifatturiero, lo sapete, signori del Governo; lì c'è il nerbo della nostra capacità competitiva. Voi avete cominciato a rispondere al drammatico problema propostoci da quei dati con un taglio della spesa in conto capitale del 20 per cento tra il 2009 e il 2008: non è mai stato operato un taglio di queste dimensioni nella spesa in conto capitale nella storia della Repubblica italiana! Avete risposto con l'eliminazione dei residui crediti d'imposta automatici sopravvissuti alla falcidie (sempre vostra) nel 2002. Immorali, ha detto a proposito dei crediti d'imposta automatici il Ministro, perché darebbero luogo ad abusi. È uno strano modo di ragionare: in contrasto con i principi elementari di etica politica, cioè immorale, sembra piuttosto uno Stato che penalizza tutti gli onesti perché non sa individuare e colpire per tempo i farabutti. Tra pochi giorni saranno pubblicati i dati dell'ISTAT sull'occupazione dell'ultimo trimestre, il primo della crisi. Vorrei tanto sbagliarmi, lo dico sinceramente, ma credo che ci parleranno della già avvenuta distruzione di qualche decina di migliaia di posti di lavoro, più di quanti - prevedo - ne distrusse nei primi tre mesi la crisi del 1992-1993, che alla fine ne eliminò quasi un milione, non dimentichiamocelo. Davvero pensate che basti, signor Ministro, rispondere con la concessione della cassa integrazione in deroga? Anche voi sapete

E sapete che i contenuti non ci sono non perché siete cattivi o perché non volete metterceli, ma perché per esserci i contenuti reclamano risorse aggiuntive, che a loro volta non ci sono perché voi non volete cambiare il segno della vostra politica di bilancio, da duramente restrittiva a responsabilmente espansiva. Il ragionamento torna così alla domanda iniziale: perché questa politica di bilancio così ottusa? E fornisce la risposta giusta, finalmente: voi non cambiate politica fiscale non perché non sapete che sarebbe necessario, ma perché sapete benissimo di non avere la forza politica necessaria per attuare questa svolta, perché alla fine dei conti la vostra è una coalizione di forze ancora dotata di grandissimo consenso, lo sappiamo, ma nella quale prevale un orientamento conservativo, mentre è il cambiamento in tutti i campi la leva che ci può sollevare oltre la crisi, quel cambiamento che noi vi abbiamo proposto e che voi avete rifiutato. Votiamo contro con animo sereno, lasciandovi piena la responsabilità di questa scelta destinata ad essere pagata duramente dal Paese e dalla componente più debole del nostro popolo.

Signor Presidente, colleghi senatrici e senatori, stiamo per approvare la legge finanziaria 2009. Conosciamo benissimo il contesto internazionale in cui essa si è sviluppata, un contesto caratterizzato da una crisi gravissima, una crisi gravissima, per tanti versi inedita, nella quale l'Italia si è trovata in una posizione abbastanza dissimile anche da altri Paesi europei. Ad esempio, l'Italia si è venuta a trovare in una situazione meno esposta ai mercati finanziari di tutti gli altri Paesi europei.

enormi quantità di capitali per consentire la liquidità del sistema finanziario. Questo significa che abbiamo dei fondamenti, almeno sul piano finanziario, più sani e meglio strutturati di altri Paesi. Non c'è dubbio che ciò è dovuto anche, naturalmente, ad una certa impostazione della politica economica e finanziaria. luglio il decreto-legge n. 112 ha anticipato le misure che si rendevano necessarie per affrontare la crisi. Si può opinare sulla qualità delle stesse, ma non si può opinare sulla loro assoluta tempestività e forse anche sulla loro preveggenza.

l'Italia si sarebbe trovata, in questo autunno, in condizioni di gran lunga più difficili. Noi lo abbiamo evitato con il decreto del luglio scorso. Tutto si può fare meglio. Alcune misure si possono perfezionare e qualche altra cosa si dovrà cambiare, ma l'aver portato la Repubblica italiana in quelle condizioni nella crisi che abbiamo vissuto è stato un merito di questo Governo e di questa maggioranza. Non lo possiamo in alcun modo dimenticare. D'altra parte, era necessario agire così perché l'Italia è il Paese a maggior debito pubblico dell'Occidente in rapporto alla sua economia e questo è un problema che abbiamo molto ben presente. Perciò è stato necessario continuare, anche con queste misure e con questa finanziaria, nella politica di rigore nella finanza pubblica che abbiamo ritenuto non solo premessa indispensabile per le misure di sviluppo delle quali parlerò tra poco, ma per noi una misura indispensabile per poter rispettare i parametri europei, nonché i parametri di mercato. Tutto ciò non può che essere ascritto al merito del Governo e della maggioranza. Non solo, ma abbiamo continuato. Avevamo detto che la legge finanziaria sarebbe stata snella e attenta attenta soltanto alle grandi questioni e così è stato. E lo è stato non soltanto nel provvedimento che è uscito dal Consiglio dei ministri a settembre, ma anche nel suo cammino parlamentare. Questa è stata una novità importante che questo Governo e questa maggioranza hanno portato nella sessione di bilancio e ciò, nell'ambito del contesto europeo e internazionale, ha reso l'Italia più credibile. È un dato assolutamente ineccepibile. Non solo. Il Parlamento ha saputo interpretare lo spirito del Governo: nella sessione di bilancio al Senato sono state approvate soltanto alcune importanti misure necessarie e una di esse attiene proprio a quella finanza responsabile e attenta di cui si è parlato poc'anzi. Penso alla misura sul patto di stabilità e gli investimenti sui Comuni che, nell'ambito di un rigore nella finanza pubblica, affronta il problema dello sviluppo cercando di dare spazio agli investimenti degli enti locali e non alla spesa corrente. mi pare una misura assolutamente ineccepibile, che - ad onor del vero va detto - è stata approvata all'unanimità in Commissione quando è stata proposta; così come all'unanimità sono state approvate praticamente quasi tutte le modifiche che il Senato ha introdotto. per corroborare il senso della responsabilità che in questo caso questo ramo del Parlamento ha mostrato - ribadisco - in maniera ineccepibile e molto responsabile.

completerà il quadro di finanza pubblica anche sotto il profilo procedimentale, normativo e regolamentare. È qualcosa che stiamo per fare e che completa anche sotto questo profilo l'idea chiara che abbiamo. Mi pare insomma che in questo contesto così difficile abbiamo dato francamente una risposta non buona, ma davvero molto buona. Come al solito, tutto tutto si può perfezionare, ma in questo contesto aver tenuto la barra a dritta per i conti pubblici, aver aperto lo spiraglio per alcuni investimenti immediati, aver cominciato a programmare gli investimenti per il futuro, aver semplificato il procedimento, aver contribuito a modificare in senso positivo la normativa, aver completato questo provvedimento con le misure sullo sviluppo, con le misure sulle banche per i procedimenti finanziari (provvedimento che abbiamo approvato di recente in questa Camera), aver in animo di approvare dispositivi normativi per il bilancio, la cui revisione sarà uno strumento ineccepibile e molto forte per contenere la spesa corrente